Signor Presidente, «l'istallazione di un sistema di difesa missilistica in Europa orientale è praticamente una dichiarazione di guerra»: così ha scritto ieri sulla stampa italiana il grande intellettuale statunitense Noam Chomsky, che così ha proseguito: «Provate ad immaginare come reagirebbe l'America se la Russia, la Cina, l'Iran o qualunque potenza straniera osasse anche solo pensare di collocare un sistema di difesa missilistica sui confini degli Stati Uniti o nelle loro vicinanze, o addirittura portasse avanti questo piano. In tali inimmaginabili circostanze, una violenta reazione americana sarebbe non solo quasi certa, ma anche comprensibile e ciò perché» - prosegue Chomsky - «è universalmente noto che la difesa missilistica è un'arma di primo colpo». Che cos'è, dunque, questo pericolosissimo e nefasto scudo missilistico statunitense che dovrà essere installato in Europa e che il Governo italiano sembra aver accettato e segretamente concordato con la Casa Bianca? Perché, di fronte ad una questione di così grande dimensione strategica, il Parlamento italiano non è stato messo - e non è ancora messo - in condizione di discutere e decidere autonomamente? Perché tale questione non la si rende di pubblico dominio? Perché non la si racconta al nostro popolo? Volevo solo, signor Presidente, ricordarle un dato: nella Repubblica Ceca, Paese coinvolto nel progetto USA di scudo missilistico, il movimento pacifista, le forze democratiche e i giovani comunisti hanno già raccolto 300.000 firme, volte ad ottenere un *referendum* sulla collocazione dello scudo stellare. Una grande mobilitazione sociale che ha contribuito alla messa fuorilegge dei giovani comunisti cechi. È questo il prezzo che i popoli europei dovranno pagare per il progetto americano? E cioè: subordinazione alle politiche di guerra di Bush, allineamento, sottomissione delle volontà popolari e svuotamento dei poteri parlamentari? Ma che cos'è, nel concreto, lo «scudo stellare europeo»? Il piano statunitense prevede l'installazione dei primi 10 missili intercettori in Polonia e di una stazione radar nella Repubblica Ceca. La funzione dei missili intercettori è distruggere i missili balistici nemici una volta lanciati. Sul territorio statunitense ne sono già stati installati 17, di cui 14 in Alaska e 3 in California, che saliranno a 21 nel 2007 e a 30 nel 2008. Nel momento in cui gli Stati Uniti porteranno a termine lo "scudo" anti-missili disporrebbero di un sistema non di difesa, ma di offesa: sarebbero infatti in grado di lanciare una *first strike* contro un Paese dotato anch'esso di armi nucleari, fidando sulla capacità dello scudo di neutralizzare o attenuare gli effetti di un'eventuale rappresaglia. Proprio per questo USA e URSS avevano stipulato nel 1972 il Trattato ABM volto a proibire tali sistemi e che l'Amministrazione Bush, significativamente, ha cancellato nel 2002. Ufficialmente, l'installazione dei missili intercettori in Europa dovrebbe servire a proteggere gli Stati Uniti e l'Europa stessa dai missili balistici della Corea del Nord e dell'Iran. Nessuno di questi Paesi, né un altro «Stato canaglia», ha però oggi missili in grado di minacciare gli Stati Uniti e l'Europa. Per di più, la Corea del Nord, se volesse colpire gli Stati Uniti, lancerebbe i suoi missili non certo verso ovest e al di sopra dell'Europa. E se si volessero neutralizzare i missili iraniani, che non possono raggiungere gli USA e l'Europa, né sono armati di testate nucleari, occorrerebbe installare i missili intercettori in Turchia o in altri Paesi limitrofi. Secondo Mosca, il piano statunitense di installare missili intercettori nell'Europa orientale mira, essenzialmente, ad acquisire un ulteriore vantaggio strategico sulla Russia ed è per questo che al Pentagono pensano di installare altri missili ancora più a est, probabilmente in Ucraina. Allo stesso tempo potrebbe essere aumentata la loro gittata, così da minacciare i sistemi spaziali russi, né può essere sottovalutata la possibilità che questi missili siano un giorno armati di testate nucleari. Immediato è il vantaggio che gli USA possono acquisire installando in Europa stazioni radar analoghe a quella che intendono collocare nella Repubblica Ceca. Essa sarebbe la prima installazione di una rete di sofisticati centri di *intelligence*, attraverso cui il Pentagono potrebbe monitorare, ancor più più efficacemente di quanto è in grado di fare oggi, non solo il territorio russo, ma l'intero territorio europeo. L'Italia, per la sua posizione geografica, sarebbe inoltre particolarmente adatta per l'installazione sia di radar che di missili intercettori rivolti verso il Medio Oriente e il Nord Africa. L'altro vantaggio per Washington sarebbe quello di avere in mano un altro strumento per impedire che l'Unione Europea possa un giorno rendersi militarmente autonoma dagli Stati Uniti. L'intero sistema di stazioni radar e postazioni missilistiche in Europa dipenderebbe infatti dal Centro di comando, controllo, gestione della battaglia e comunicazioni, all'interno della catena di comando che fa capo al Presidente degli Stati Uniti d'America. È dunque facile capire - tra l'altro - che sul piano geopolitico uno degli obiettivi primari dell'installazione dello scudo americano è la divisione chirurgica dell'Europa: da una parte l'area originaria dell'Unione Europea, dall'altra un'Europa dell'Est, sottomessa politicamente, economicamente e militarmente agli USA con due obiettivi: l'interruzione del progetto di costruzione di una grande Europa, pericolosa per gli USA, e la messa in campo di un vasto fronte specificamente militare contro la Russia. La Russia, di fronte al tentativo statunitense di acquisire un ulteriore vantaggio strategico nei suoi confronti, ha già annunciato che prenderà delle contromisure, adottando «metodi adeguati e asimmetrici» e Putin ha già annunciato la moratoria del Trattato sulle Forze armate convenzionali in Europa, firmato dai Paesi della NATO e del Patto di Varsavia nel 1990. Il piano statunitense di installare missili intercettori e radar nell'Europa orientale, a ridosso del territorio russo, viene dunque considerato a Mosca un ulteriore passo dell'espansione della NATO ad est. La risposta di Putin al progetto di scudo stellare è stata durissima ha evocato tutto il pericolo insito nella scelta americana: Putin ha avvertito che se gli Usa installeranno missili e radar a ridosso del territorio russo, la Russia potrebbe anche ritirarsi dal Trattato INF del 1987, che ha permesso di eliminare i missili nucleari a raggio intermedio in Europa. L'Europa, e in particolare l'Italia, che ha già aderito al programma dello scudo statunitense, rischia di ricadere nell'incubo politico e militare di una nuova guerra fredda che ha buone possibilità di trasformarsi in una guerra nucleare. L'Accordo quadro prevede una serie di accordi specifici che coinvolgeranno nel programma dello "scudo" statunitense non solo le industrie militari italiane, soprattutto quelle del settore aerospaziale, ma anche università e centri di ricerca. L'accordo quadro comporta, quindi, un'ulteriore militarizzazione della ricerca, a scapito di quella civile, sotto la cappa del segreto militare. Comporta un ulteriore aumento della spesa militare italiana (già al settimo posto su scala mondiale), soprattutto dei programmi di investimento derivanti da accordi internazionali, ai quali l'ultima finanziaria ha destinato 4,5 miliardi di euro in tre anni. Comporta un ulteriore rafforzamento dei comandi e delle basi statunitensi in Italia, comprese quelle dotate di armi nucleari, con la conseguenza che il nostro Paese diverrà ancor più trampolino di lancio delle operazioni militari statunitensi verso Sud e verso Est. Comporta ulteriori pericoli per il nostro Paese, che, per la sua collocazione geografica, costituisce una postazione ottimale in cui installare i missili intercettori: le zone di installazione diverranno di conseguenza bersagli militari, come negli anni Ottanta la base di Comiso, in cui erano installati i missili nucleari statunitensi. Inoltre, estendendo lo «scudo» all'Europa, gli USA potrebbero scaricare sugli alleati parte dei costi per lo sviluppo del sistema, ammontanti finora a 10 miliardi di dollari annui. In questo quadro estremamente pericoloso, appare appare davvero inquietante il comportamento del Governo italiano, particolarmente reticente nel raccontare i fatti relativi all'accordo con il Governo statunitense sullo «scudo stellare» e i fatti relativi alla firma dell'accordo. Il generale Henry Obering, direttore dell'Agenzia USA di difesa missilistica, ha annunciato il 27 marzo 2007, di fronte al Comitato per i servizi armati della Camera dei rappresentanti, che l'Italia entra ufficialmente nel programma dello «scudo» antimissile che gli Stati Uniti vogliono estendere all'Europa. «Ho il piacere di annunciare che lo scorso febbraio abbiamo stabilito un *memorandum* di Accordo quadro con l'Italia e possiamo ora iniziare a sviluppare possibilità di condivisione, tecnologie di difesa missilistica, analisi, e altre forme di collaborazione». Così ha parlato il generale americano Henry Obering. Nessun annuncio, invece, da parte del Governo italiano. Quando il 12 marzo il segretario generale della NATO Jaap de Hoop Scheffer dichiara che «in materia di difesa missilistica non ci devono essere Paesi di «serie A» e Paesi di «serie B» all'interno della NATO», il ministro degli esteri Massimo D'Alema dice di condividere l'opinione di Scheffer, auspicando che la proposta degli Stati Uniti di estendere il loro «scudo» all'Europa venga discussa dalla NATO e dall'Unione Europea. Non dice, però, che l'Italia ha, a questo punto, già sottoscritto il *memorandum* di Accordo quadro ed è stata quindi promossa in «serie A». La firma dell'Accordo quadro viene dunque tenuta segreta al Parlamento e, a quanto si dice, anche a parte della coalizione governativa. Il Governo italiano ha anche smentito, dobbiamo dire un po' affannosamente, di aver firmato l'accordo con il Governo USA. Ma le contraddizioni all'interno del Governo sono davvero strane e, per certi versi, sconcertanti. Il sottosegretario di stato alla difesa Marco Verzaschi, dell'Udeur, ha infatti dichiarato, il 12 aprile 2007 alla Camera dei deputati: «Da parte italiana, è stato recentemente firmato un Accordo quadro di cooperazione Italia-USA che amplia il perimetro di tale cooperazione al settore della difesa da missili balistici». Il sottosegretario Verzaschi non ha però spiegato non ha però spiegato perché il Governo italiano avesse finora tenuto segreto un accordo di tale portata, né ha precisato chi l'abbia firmato lo scorso febbraio. Il sottosegretario alla difesa Giovanni Forcieri aveva annunciato, tramite la sua segreteria, che avrebbe ufficialmente smentito di averlo firmato lui. A ciò che ci risulta, però, il sottosegretario Forcieri deve ancora far pervenire la propria smentita. L'accordo per lo «scudo» sarebbe avvenuto, dunque, in ambito NATO, come dicono alcuni, tra cui lo stesso Verzaschi? Non sembra affatto di questo parere il generale Obering, che ha invece chiarito che lo schieramento in Europa, da parte degli Stati uniti, di missili anti-missili non rientra in ambito NATO e che «gli USA non sono disponibili a cedere la responsabilità del progetto». Le ultime elezioni amministrative, signor Presidente, ci dicono chiaramente che il Governo Prodi rischia di consumare il rapporto con il proprio blocco sociale di riferimento. La fiducia nei confronti del Governo Prodi si va riducendo giorno dopo giorno. Non potremo certo riconquistarla proseguendo politiche di guerra al servizio della potenza americana, né, tanto meno, spostando enormi risorse economiche dalla spesa sociale a quella militare. Vi sarebbe una sola parola d'ordine per costruire l'alternativa e ridare fiducia al nostro popolo: via dall'Afghanistan e via dalle guerre, più autonomia dagli Stati Uniti e dalla NATO, meno favori alle grandi fortune capitalistiche e, finalmente, più Stato sociale, più salari

in una *querelle* internazionale molto ampia, che riguarda un accordo bilaterale tra Stati Uniti, Repubblica Ceca e Polonia circa l'installazione di radar e rampe missilistiche, che ha molto irritato - ed è un eufemismo - la Russia. Si tratta del programma *Ballistic* *Missile* *Defense* *System*, che prevede l'installazione di missili intercettori la cui funzione è di distruggere missili balistici nemici una volta intercettati.

trattato ABM, già affossato dall'Amministrazione Bush nel 2002. Le reazioni della Russia non sono tardate, aumentando una ripresa dell'*escalation* militare che alimenta un clima da vera e propria guerra fredda.

Questo scontro sull'installazione del sistema antimissile ha determinato reazioni forti anche in Europa (abbiamo sentito le dichiarazioni di Solana, della Merkel e di Chirac) che, al di là del merito, criticavano fortemente il metodo degli accordi bilaterali stipulati al di fuori dell'Unione Europea e in subordine stipulati nella NATO. Il ministro D'Alema ha affermato in quell'occasione che la discussione sul sistema di difesa dei missili balistici è partita male perché posta in ambito bilaterale. Dichiarazione condivisibile, ma in parte sorprendente - su questo vorrei che il Sottosegretario mi rispondesse - perché, quando il Ministro l'ha pronunciata, l'Italia aveva già firmato un Accordo bilaterale con gli Stati Uniti per la cooperazione nel settore della difesa da missili balistici e questo in segreto (lo diceva il collega), al di fuori di un voto o di un'informazione non solo al Parlamento - ed è già grave ma persino al Consiglio dei ministri. In base a questo accordo, segreto in Italia, ma reso noto dal generale Obering (responsabile dell'Agenzia missilistica del Pentagono) in un'audizione al Senato americano (e arrivo all'oggetto della mia interpellanza), aziende di aziende di Finmecanica (ELSAG-Datamat) si sono già aggiudicate l'incarico di realizzare componenti del *Ballistic System*, nella fattispecie *software*. E infatti il ministro D'Alema ha dichiarato:

tecnica e non perturbante per le relazioni internazionali. Quindi, da una parte si critica - ed è giusto - il metodo bilaterale, anche se è esattamente quello che abbiamo seguito noi; dall'altra, si minimalizza a parole la partecipazione al progetto dei missili balistici, facendolo passare per una mera cooperazione tecnologica, interessante dal punto di vista industriale, che, lo sappiamo bene, è il modo per rendere sostanziale e potenzialmente irreversibile - è sempre così e il sottosegretario Forcieri lo sa meglio di me la cooperazione politica al progetto e al futuro finanziamento (che adesso non c'è, come ha detto anche il sottosegretario Verzaschi). Accordo che anche per il momento non si limita ad uno scambio di informazioni, ma, in modo analogo agli Accordi firmati da altri Paesi sullo stesso progetto, è l'anticamera della partecipazione attiva complessiva al progetto *Ballistic* *Missile* *Defense* *System*. Molti Paesi che hanno firmato inizialmente un accordo quadro di massima adesso vi partecipano in modo attivo:

il Giappone con navi e radar, Israele con missili a intercettazione terminale. Insomma, queste le dichiarazioni di Obering. Allora, considerate le negative avvisaglie internazionali che alimentano la guerra fredda (diciamolo,

Russia come minaccia); considerato che le intercettazioni previste da questo sistema costituirebbero un pericolo anche per le popolazioni europee e un mutamento degli equilibri in atto; considerato che, comunque, i centri di comando e di controllo di questo sistema che impartiscono gli ordini di lancio dei missili schierati in Europa si troverebbero e si trovano sempre e solo negli Stati Uniti; considerato che il segretario generale della NATO, De Hoop Scheffer, ha affermato che il tema vero è intercettare le traiettorie dei paventati missili iraniani e, quindi, occorrerà ampliare il cosiddetto scudo all'area mediterranea, che è una promessa e una minaccia al tempo stesso; considerato che il ministro D'Alema ritiene «auspicabile questo sistema di difesa», anche se pensa

che un sistema di difesa antimissile è vietato - l'ho detto all'inizio, la ritengo una cosa grave - dal Trattato ABM e costituisce un passo nella direzione della guerra fredda,

importanza effettuate nelle segrete stanze per tenere all'oscuro non solo l'opinione pubblica, ma anche il Parlamento. Tutto ciò è assolutamente illegale e vietato dalla Costituzione e dalle leggi. Basti pensare che le bozze degli Accordi internazionali devono essere presentate e discusse nel Consiglio dei ministri e gli stessi accordi devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. I quesiti sembrano quasi minimali rispetto a questa premessa allarmata; sapere se il Ministro non ritenga di dover far conoscere questo programma. La collega Deiana, alla Camera dei deputati, lo ha chiesto e tuttora rimane segreto; noi, in Commissione difesa, al Senato, abbiamo chiesto di conoscerlo

infatti tanti nomi e, secondo me, è giusto sapere chi lo ha firmato e in base a quali motivazioni e autorizzazioni. Riteniamo inoltre che, alla luce delle valutazioni espresse anche da alti esponenti dell'Unione Europea, la partecipazione senza previa concertazione con i *partner* europei in una materia così rilevante sul piano dei rapporti internazionali e così disequilibrante rispetto alla Russia, costituisca un'oggettiva frattura all'interno dell'Europa e un pericolosissimo precedente.

le considerazioni che sono state svolte, al di là di alcuni eccessi di valutazione anche verbali, potrebbero avere un fondamento se

pensare di poter compiere in una materia così delicata degli atti segreti che non vengono sottoposti all'attenzione del Parlamento e dell'opinione pubblica; direi, tuttavia, che questa descrizione non corrisponde alla realtà dei fatti. Cercherò di rispondere congiuntamente alle due interpellanze perché si tratta di di materia attinente e mi auguro di poter riuscire a dare informazioni che possano sgombrare il campo da quelle preoccupazioni che gli interpellanti hanno espresso nella loro illustrazione. Vorrei anch'io ricordare che sul tema il Governo ha già risposto alla Camera dei deputati in due occasioni, il 22 marzo e il

ha recentemente firmato un Accordo quadro di cooperazione Italia-USA nel settore della difesa da missili balistici e non (voglio sottolineare il «non»), un accordo sul cosiddetto scudo antimissili, così com'è stato paventato. Tale Accordo quadro di cooperazione, firmato il 16 febbraio 2007 dal Ministro della difesa, si inserisce nelle molteplici iniziative intraprese in ambito NATO dove, fin dal 1996, sono state avviate varie attività volte alla realizzazione di idonei strumenti a protezione dell'Alleanza dal rischio derivante dall'uso di missili balistici equipaggiati con armi di distruzione di massa da parte di Nazioni ostili o di gruppi terroristici. L'Accordo in questione muove dalla volontà dei due Paesi di creare un quadro normativo di riferimento che consenta alle due Nazioni di rafforzare la cooperazione in ambito bilaterale in tale specifico settore, per consentire di dare l'avvio a scambi di informazioni.

In particolare, per l'Italia appare necessario avviare uno scambio di informazioni per supportare lo sviluppo di una *policy* nazionale, basandosi sulle attività in corso negli Stati Uniti con il programma di difesa del territorio e della popolazione da missili balistici, denominato - com'è già stato ricordato - «*Ballistic* *Missile Defense System*» e in vista della possibilità che la NATO decida di dotarsi di un sistema similare in grado di difendere territori e popolazioni dell'Alleanza, così come in sede NATO si sta da tempo discutendo. Senatrice

(*Active Layered Theatre Ballistic Missile Defense*) che ha lo scopo di sviluppare un sistema per la protezione di forze di teatro contro missili di breve gittata.

generale che consenta agli Stati di contribuire con i sistemi che hanno già a disposizione: quindi, la messa in comune dei sistemi già a disposizione che possa consentire la protezione delle truppe in teatro. in teatro. C'è poi il progetto citato degli Stati Uniti per la difesa territoriale di quella Nazione e c'è un programma NATO, denominato «*Missile Defense*», che tende alla realizzazione di un sistema di protezione per i territori delle Nazioni NATO. Questo è uno degli argomenti ancora in discussione, sia dal punto di vista dei princìpi generali e ancor di più nel merito della sua attuazione. Recentemente, gli Stati Uniti

In tale ambito, per quanto riguarda la notizia riportata dal quotidiano «Il Secolo XIX», citata dall'interpellanza della senatrice Pisa, si deve precisare innanzitutto che nessuna impresa nazionale è impegnata nel progetto,

quello per la protezione delle forze sul teatro, che non ha alcuna connessione o attinenza con il il citato BMDS e che non ha niente a che vedere con l'accordo quadro citato, di cui stiamo discutendo, firmato tra gli Stati Uniti e il nostro Paese. L'accordo firmato, inoltre, non comportando impegni attuativi specifici né oneri finanziari, ma avendo solo lo scopo di definire un *framework* legale per un preliminare scambio di informazioni in tema di difesa missilistica e di individuare possibilità/modalità di impegno delle parti nell'ambito della ricerca e sviluppo, non necessitava, ai fini della sua sottoscrizione, del preventivo parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Questa è stata la valutazione fatta, avendo queste caratteristiche l'accordo. Quanto alla difesa missilistica, in realtà essa si inquadra nel più generale concetto di deterrenza e prende spunto dalla natura imprevedibile ed asimmetrica delle nuove minacce provenienti dal terrorismo internazionale e, come ho detto prima, dagli Stati potenzialmente ostili, proliferatori di armi di distruzione di massa. È in questo quadro - dicevo - che si collocano i programmi portati avanti in ambito NATO e quelli sviluppati sul piano bilaterale con gli Stati Uniti da alcuni Paesi europei: li avete citati voi, tali Paesi, e certo il nostro non fa parte di questo tipo di accordi. Infatti, l'amministrazione americana ha dato nuovo slancio ai programmi nazionali di difesa missilistica, come dicevo prima. prima. Sapete che sono state previste la postazione di radar sia in Alaska che in California e adesso la postazione per la Repubblica Ceca e per la Polonia. Ilprogetto che, come ho detto, era stato inizialmente concepito in funzione della difesa nazionale, potrebbe essere evoluto a programma volto a tutelare anche i territori e le popolazioni dei Paesi alleati ed amici. Infatti, i principali alleati degli Stati Uniti sono stati incoraggiati ad associarsi ai progetti americani e sono state avviate cooperazioni, oltre che quella nei termini come ho descritto prima con il nostro Paese, anche con altri Paesi tra i quali il Giappone, il Regno Unito, la Danimarca, l'Australia, Israele, l'Olanda e la Russia. Ha citato la senatrice Pisa il fatto che alcuni di questi Paesi hanno poi proseguito la loro cooperazione e collaborazione, andando avanti anche nel partecipare più pienamente a questo sistema: è una decisione è una decisione autonoma presa da quei Paesi, che non può essere presa minimamente a riferimento per decisioni del nostro Paese, che non ha intenzione di procedere in questa direzione. Peraltro, la difesa contro la proliferazione della minaccia missilistica è avvertita in seno all'Alleanza atlantica come un'esigenza preminentemente protettiva, anche se al riguardo ci sono interpretazioni. Abbiamo tutto letto ieri su «il manifesto»

quanto riguarda, invece, la questione citata nell'interpellanza in merito alla ricaduta di detriti radioattivi, credo sia giusto far notare che questo è ancora uno dei temi in discussione, ad esempio nell'ambito NATO, e che comunque il sistema tenderebbe a colpire nello spazio in modo da disintegrare direttamente o poi con il passaggio in atmosfera qualsiasi tipo di frammento. Naturalmente questo è un obiettivo. Non è detto che finora si sia raggiunto. È giusto che sia un tema di discussione e lo è attualmente in ambito all'Alleanzaatlantica. Ciò posto, da un punto di vista tecnico non avrei altro da aggiungere. Passando al quadro delle alleanze e della politica estera del nostro Paese che sono state citate dagli interpellanti, che riguardano la questione in esame, si osserva che anche in ambito NATO esistono avanzati programmi di cooperazione che mirano alla protezione di tutti i territori e delle popolazioni alleate. È fuor di dubbio che la difesa missilistica abbia - come detto - una finalità protettiva, ma nuovi programmi sono, comunque, suscettibili di alterare equilibri strategici consolidati, in particolare con la Russia. Di questo il nostro Paese ne è convinto e ne è preoccupato. Infatti, il Ministro degli affari esteri dell'Italia, unitamente ad esponenti di altri Paesi *partner* europei, tra i quali il Primo ministro tedesco, ha convenuto sull'opportunità che tale materia sia affrontata in ambito NATO, quindi in un ambito multilaterale e non in ambiti bilaterali, anche nel formato NRC (cioè del Consiglio NATO-Russia), così come anche nella dimensione dell'Unione Europea. Il Governo americano ha, peraltro, più volte sottolineato, sia nell'ambito dell'Alleanza atlantica, che nel corso di contatti bilaterali con la Russia, le finalità prettamente difensive di tali sistemi, collegandole espressamente ed esclusivamente a potenziali minacce provenienti dal quadrante orientale e mediorientale. Nelle ultime settimane, poi, anche da parte americana è stata manifestata ampia disponibilità ad inserire a pieno titolo la difesa missilistica tra le questioni in discussione nel quadro del Consiglio NATO-Russia. L'Italia auspica che questo confronto possa continuare ed anzi rafforzarsi, in uno spirito costruttivo e senza preclusioni pregiudiziali, poiché esso valorizza il ruolo di strumento di dialogo politico del Consiglio NATO-Russia, soprattutto in materia di sicurezza. Esso, inoltre, giova a dissipare i timori da parte di Mosca, che meritano, tuttavia, di essere tenuti in debita considerazione e riscontrati. L'Italia è da sempre, con coerenza, impegnata in tutti i fori nella promozione degli strumenti multilaterali di non proliferazione, controllo degli armamenti e disarmo e nella ricerca di soluzioni pacifiche e negoziali delle controversie internazionali; aspetti, questi, che costituiscono un caposaldo della politica estera del nostro Governo e anche della politica di difesa e di sicurezza. Anche nel corso della riunione informale dei Ministri degli esteri tenutasi di recente a Oslo, il ministro D'Alema ha avuto modo di ribadire la nostra posizione, peraltro largamente condivisa, che è riassumibile nel modo seguente. l'Italia giudica seria la minaccia della proliferazione missilistica e attribuisce importanza all'approfondimento delle possibili opzioni di difesa per l'Alleanza. altresì apprezzato ed incoraggiato l'approccio costruttivo e la trasparenza che hanno caratterizzato sinora le consultazioni NATO in materia di difesa missilistica, con particolare riguardo alle installazioni in Europa previste dall'estensione del programma nazionale americano. Le consultazioni intercorse hanno messo in luce l'impegno degli Stati Uniti per fugare le preoccupazioni degli alleati in merito alla indivisibilità della sicurezza euroatlantica e della Russia in relazione agli equilibri strategici. Siamo anche noi contrari al fatto che possano essere che possano essere considerati alcuni alleati di serie A, altri alleati di serie B. In secondo luogo, tenendo a mente il principio della indivisibilità della sicurezza della NATO, l'Italia appoggia con convinzione il lavoro già avviato dal Consiglio atlantico stesso, inteso a raccordare gli attuali programmi comuni di difesa missilistica e quelli nazionali, tra cui quello americano. In terzo luogo, viene, altresì, attribuita estrema importanza alla prosecuzione di un dialogo franco e costruttivo con la Russia in questo campo, dialogo che, oltre ad accrescere la reciproca trasparenza e fiducia, è suscettibile di dischiudere nuovi, importanti spazi di cooperazione, di cooperazione, al di là dell'attuale quadro di attività comune sui missili di teatro. A questo proposito, credo che non ci siano alternative allo sviluppo di un rapporto positivo dell'Unione Europea con la Russia, superando anche alcuni eccessi che alcuni Paesi dell'Unione Europea hanno manifestato nei confronti di questo importante *partner*, che per il nostro Paese è di natura prioritaria. Il dibattito che si è tenuto nel corso delle ultime settimane sulla difesa antimissile ha dimostrato, ancora una volta, il valore strategico del Consiglio NATO-Russia, appunto, e la sua capacità di attenuare tensioni e incomprensioni e di trasformare questioni controverse in materia di cooperazione. Nel prossimo mese ci sarà un importante riunione di questo organismo con l'intero Consiglio Atlantico (a celebrazione del X anniversario della sua costituzione e del quinto anniversario

Rispondendo, quindi, a uno dei quesiti formulati dai senatori interpellanti, non si ravvedono profili di contrasto tra le recenti posizioni espresse dal ministro degli affari esteri, onorevole D'Alema, e l'accordo quadro di cooperazione USA-Italia di cui si è parlato. In conclusione, l'Accordo quadro in questione rappresenta lo strumento normativo che consente al nostro Paese di ampliare la cooperazione con gli Stati Uniti anche nel settore della difesa da missili balistici, al fine - ripeto - di consentire uno scambio informativo nello specifico settore, nella prospettiva delle discussioni in sede NATO, lasciando del tutto impregiudicate eventuali decisioni future che, con quest'atto, non sono minimamente compromesse e tanto meno pregiudicate.

Onorevoli colleghi, la notte del 10 agosto la ricordiamo come la notte di San Lorenzo e del suo martirio. Racconta la leggenda che lui ha pianto e ha fatto scorrere copiose lacrime; queste lacrime, con un atto di bontà della divina previdenza, si sono trasformate in stelle cadenti. È per questo che ogni 10 agosto i bambini guardano il cielo gioiosi, perché possono vedere le stelle cadenti. Cosa fate voi del Governo e noi di questo Parlamento? Vogliamo trasformare le illusioni magiche ancora una volta nella percezione del pericolo reale che il cielo possa costellarsi di luci di missili? Signor Sottosegretario, le agenzie, alle ore 14,46 di oggi, 31 maggio, riportano una durissima dichiarazione del presidente Putin, in cui «Gli americani hanno abbandonato il Trattato ABM. Li abbiamo avvisati che a nostra volta avremmo prodotto una risposta per mantenere un equilibrio strategico nel mondo. Non abbiamo cominciato noi» - ha insistito Putin - «ma questa è una nuova corsa agli armamenti». Questa dichiarazione Questa dichiarazione è decisiva. Non siamo soddisfatti, signor Sottosegretario. Non serve dire che il nostro Ministero degli affari esteri si impegnerà in un rapporto costruttivo con la Repubblica russa. Il dato concreto è questo: la Repubblica russa ha dato la sua risposta. Noi chiediamo un ampio e chiaro dibattito, senza segreti militari, senza giochi di parole sulla questione del coinvolgimento dell'Italia, sia in forma diretta che indiretta, nella questione chiamata scudo missilistico. Noi chiediamo che l'Italia non partecipi a questa scalata militaristica, che non ci tuffi in questo girone infernale che potrà oggettivamente compromettere la vita nostra e delle future generazioni.

e tengo molto al Governo dell'Unione, ma proprio perché ci tengo pretendo verità e trasparenza. Sul resto

che ha votato e dato fiducia al Governo e che è stato ripagato con il raddoppio delle spese per gli armamenti, nonostante il programma dell'Unione prevedesse la riduzione delle spese degli armamenti, che è stato ripagato con il raddoppio e l'ampliamento della base di Vicenza, nonostante il programma dell'Unione prevedesse la rinegoziazione. trova di fronte a questo accordo che viola persino trattati internazionali come il trattato ABM. Allora, credo che siamo di fronte ad una delusione. Il nostro popolo è molto grande e vorrei tanto che non continuassimo a farci del male

in relazione all'interrogazione del senatore Gramazio è opportuno ricordare che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della legge 14 aprile 1975, n. 103, non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte concernente la programmazione televisiva. Come è noto, infatti, la menzionata legge ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'attività governativa per assegnarla alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale determina gli indirizzi dei vari programmi vigilando sul contenuto degli stessi ed adottando, qualora se ne manifesti la necessità, le deliberazioni ritenute necessarie ai fini dell'osservanza degli indirizzi medesimi. Da parte sua, il direttore generale della società concessionaria del servizio pubblico del servizio pubblico radiotelevisivo - ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 206 del 1993 - è tenuto ad assicurare, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio di amministrazione della medesima società. Ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda la *fiction* «L'ultimo dei Corleonesi» andata in onda il giorno 14 febbraio ultimo scorso, giudicata dall'onorevole senatore interrogante una «invenzione» e una «finzione» ed in merito alla quale il procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso, aveva espresso rammarico perché perché nel film era stato dato poco spazio a tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine che avevano contribuito alla cattura del pericoloso latitante protagonista della *fiction* in esame, la concessionaria RAI, sentita al riguardo, ha osservato che lo stesso procuratore citato nell'atto parlamentare cui si risponde ha avuto modo di precisare - in una dichiarazione resa all'ANSA il 13 febbraio ultimo scorso che il suo giudizio, peraltro riportato in modo preciso da alcuni quotidiani, non voleva essere una critica alla correttezza del film o alla RAI alla quale, anzi, il citato magistrato ha riconosciuto il merito di aver riportato l'attenzione generale sui temi quali la mafia e la lotta alla stessa, come dimostrato dalla programmazione, in tempi recenti, del film su Giovanni Falcone, di quello sulla storia di Padre Puglisi, della *fiction* su Provenzano, nonché della «*docufiction*» sulla cattura di quest'ultimo *boss*. Del resto - ha concluso la RAI - il medesimo procuratore, con il riferimento alla *fiction*: «mi sono più volte detto che è una *fiction*», come riportato dallo stesso onorevole senatore interrogante, ha ben sintetizzato il senso di questa, come di ogni altra rappresentazione cinematografica, che, senza nulla togliere alla verità dei fatti rappresentati, necessariamente enfatizza alcune circostanze ed alcuni personaggi, lasciandone più in ombra altri, per favorire la narrazione scenica che, in quanto tale, non può assumere i connotati

per difendere la sua posizione. Ma tornando all'interrogazione e al fatto che il procuratore antimafia Pietro Grasso indirizza proprio questo problema nei riguardi delle forze dell'ordine, voglio ricordare che qualche settimana fa cadeva l'anniversario dell'assassinio di Giovanni Falcone. Il Presidente del Senato

in risposta all'interrogazione si fa presente che, dagli atti in possesso della competente direzione generale del Dipartimento amministrazione penitenziaria, risulta che la gestione del personale, presso la Casa circondariale di Tolmezzo, è rispettosa della normativa vigente. Infatti, secondo quanto riferito dai competenti uffici, i disagi segnalati dal personale formano oggetto dì immediata disamina da parte del comandante di reparto e del direttore dell'istituto. Per quanto concerne, più nel dettaglio, le problematiche segnalate dal senatore Eufemi è possibile riferire che si fruisce normalmente dei riposi e che, a richiesta, ne è consentito anche il cumulo, seppur in maniera limitata, per la necessità di conciliare le esigenze personali con la qualità del servizio. Al 31 dicembre 2006 i riposi di cui fruire erano 476 per 202 unità, numero irrisorio se si tiene conto delle numerose festività del mese di dicembre 2006 e del contestuale periodo feriale. I criteri di distribuzione del lavoro straordinario stabiliti in sede di contrattazione decentrata vengono puntualmente osservati. Dal mese di agosto 2006, a seguito dell'applicazione della legge sull'indulto e della disattivazione di due reparti detentivi, il lavoro straordinario è stato dimezzato, passando dalle 2.500-2.800 ore medie mensili alle attuali 1.300-1.500, nel pieno rispetto degli accordi assunti. Per quanto attiene alla mensa di servizio, il relativo godimento avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti e non si registrano lamentele circa la qualità del servizio. In riferimento all'inasprimento dei procedimenti disciplinari si segnala, al contrario, un significativo decremento degli stessi nel corso degli anni, visto che si è passati dai 79 del 2004, ai 68 del 2005, fino ai 47 del 2006. Le più recenti informative dell'autorità giudiziaria si riferiscono, per gli aspetti di rilevanza penale, al rilevante fenomeno dell'assenteismo. Pertanto, la competente direzione generale si limita a seguire gli sviluppi degli eventuali procedimenti, prima di prendere in considerazione qualsiasi provvedimento. In relazione alla carenza di organico si comunica che la direzione generale ha adottato circa 20 provvedimenti di distacco in sedi extraregionali. Appaiono, quindi, infondate le lamentele riguardanti lo stile gestionale del direttore dell'istituto, l'attività di quest'ultimo è stata oggetto di proposta di encomio da parte dell'ufficio per l'attività ispettiva e del controllo. Deve, infine, farsi presente che le doglianze espresse dall'organizzazione sindacale OSAPP una situazione di malcontento del personale di polizia penitenziaria risultano non confermate dalla direzione della casa circondariale e dal provveditorato regionale di Padova. Presidente, sono completamente insoddisfatto per la risposta

per la complessità della questione. Non c'è da aspettarsi diversamente da parte dei direttori regionali, quindi è come se ogni rappresentanza parlasse male di se stessa. Lei ha riferito di un decremento, io invece voglio fare riferimento ai continui procedimenti giudiziari - circa 30 - disposti nei confronti del personale penitenziario, anche per malattia, come è accaduto per ben 13 persone, e che rilevano un profondo disagio in cui si trova questo istituto. Sono stati svolti procedimenti a carico della Polizia penitenziaria su denuncia dei detenuti, sempre risoltisi con la piena assoluzione degli imputati, con costi aggiuntivi a carico dell'amministrazione pubblica, quindi della collettività, in quanto i procedimenti con esito negativo implicano, su richiesta dell'imputato, il pagamento delle spese di difesa a carico della pubblica amministrazione. Non va trascurato poi che il personale del nucleo operativo svolge turni massacranti - questo non è stato detto - di 15-20 ore, senza alcuna iniziativa del comandante per lenire o cambiare la situazione. Quanto ho evidenziato è riferibile anche ad altri istituti, per esempio, del Piemonte: in altre interrogazioni ho portato i casi di Cuneo, Biella, Aosta, Asti. Sarebbe opportuno, allora, dare un segnale di discontinuità interrompendo le molteplici attività, per esempio, nel periodo estivo, così da assicurare soltanto i servizi essenziali, garantendo i diritti soggettivi i diritti soggettivi del personale della polizia penitenziaria che non vengono riconosciuti. In altre interrogazioni ho posto anche la necessità di intervenire con ispezioni, che non hanno avuto seguito né a livello parlamentare, né da parte del Governo, né nelle sedi preposte del capo del Dipartimento e dell'ufficio ispettivo del Dipartimento, in quanto, nonostante la presenza di personale appartenente al ruolo dei soprintendenti, la sorveglianza interna e generale viene demandata al personale appartenente al ruolo degli assistenti, in netta violazione dell'articolo 21 del regolamento del Corpo di polizia penitenziaria. inoltre una strutturale carenza di organico aggravata dalla scelta di assegnare il personale di Polizia penitenziaria a compiti non istituzionali, destinandoli ad uffici che spetterebbero al personale del comparto dei Ministeri, per esempio.